L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della salute sulla contaminazione da diossina di uova e carni». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro della salute, professor Fazio.

non vi è rischio per la salute del consumatore italiano per la presenza di diossina in uova e carne. La normativa comunitaria stabilisce quali valori massimi di diossina siano ammessi negli alimenti. Questi valori massimi sono stabiliti, in base al consumo medio dei cittadini comunitari, in picogrammi per grammo di grasso e sono pari ad un picogrammo per grammo di grasso, per la carne suina, e a tre picogrammi, per le carni bovine. Teniamo presente che in Italia i consumi medi di carne suina sono inferiori rispetto alla media della comunitaria, se i valori massimi fossero basati sul consumo italiano sarebbero evidentemente superiori. I criteri con cui vengono stabiliti i valori massimi sono molto conservativi, in termini tossicologici,

risultati positivi, per presenza di diossina, solo 24 campioni di uova, su 110 analizzati, e 2 campioni di carne di pollame, su 43 analizzati. I due campioni di carne di pollame provengono però da allevamenti bloccati, dunque, non sono mai entrati nella catena alimentare. Vorrei chiarire che i valori del campione di carne suina (l'unico risultato positivo)

Quindi, è abbastanza intuitivo che per modificare in modo significativo questo carico corporeo un uomo dovrebbe ingerire centinaia di chilogrammi di carne suina contaminata che presenti livelli di

840 picogrammi di diossina, che equivale ad una assunzione di carni suine pari a 120 chili la settimana che abbiano concentrazione massima quale quella recentemente riscontrata nel campione tedesco. Questi, quindi, i numeri.

attuale. Allo stato si può concludere che non c'è alcun rischio per la salute del consumatore italiano connesso alle problematiche recentemente emerse in Germania.

il testo proposto ai Ministri e che è stato oggetto di cosiddetta mediazione non prevede - e non la prevede tuttora - la tracciabilità delle carni suine e dei prodotti derivati dal latte. Se l'Italia avesse votato a favore di quel testo le possibilità di far passare, di fatto, il concetto che è stato definito

Per quanto attiene il problema in generale dei controlli nel nostro Paese, abbiamo voluto cogliere questa occasione per mettere a punto una serie di azioni correttive sistematiche

Il primo punto riguarda la maggiore trasparenza delle attività di autocontrollo. Poiché ci sono evidenze che dimostrano che l'esito di incidenti in sicurezza alimentare dipende anche da un processo di autocontrollo non trasparente,

cioè un disegno di legge) per assicurare che i dati generati dall'autocontrollo siano a disposizione delle autorità sanitarie in maniera fruibile e trasparente, in un sistema informatizzato accessibile non solo al Ministero ma anche alle Regioni e alle ASL.

Il secondo punto è la definizione di una netta separazione tra stabilimenti del settore alimentare e mangimistico da altri settori. Vorrei ricordare che, ancora prima che avvenisse il caso Germania, l'Italia aveva chiesto una modifica dei regolamenti

industriali) e stabilimenti alimentari e mangimistici. È noto che la ditta Harles & Jentsch produceva legalmente sia acidi grassi alimentari, sia acidi grassi destinati ad altre lavorazioni industriali, per cui poi si è verificato il noto Il terzo punto riguarda la registrazione informatizzata di tutte le imprese del settore alimentare. È intenzione di questo Governo, con le Regioni, di creare un sistema informatizzato centralizzato, alimentato su base

Il quinto punto è un incremento del 50 per cento sui controlli della sicurezza dei mangimi. In particolare, nell'ambito del Piano nazionale dell'alimentazione animale, ho disposto un aumento del 50 per cento dei campioni per la ricerca di diossina nei mangimi. Il sesto punto, che per noi ha grande rilevanza, attiene alla collaborazione con le Regioni per i siti di interesse nazionale. Posso annunciare che a breve sarà operativo (stiamo lavorando molto molto alacremente con le Regioni e le Province autonome a tal fine) un piano di monitoraggio per la ricerca dei contaminanti ambientali che hanno ripercussioni nella catena alimentare e nelle produzioni agricole in aree a rischio definite come siti di interesse nazionale, ai sensi della normativa ambientale. Questo potrebbe riguardare, per esempio, anche il noto problema di Taranto. L'ultimo punto è il piano straordinario di controllo su alimenti provenienti dalla Germania. Abbiamo disposto un piano straordinario di campionamenti *random*, ossia casuali, sugli alimenti provenienti dalla Germania. Infatti, nel rispetto del Trattato della Comunità europea, i controlli su alimenti provenienti da altri Paesi comunitari non possono essere né discriminatori né ostativi alla libera circolazione delle merci. Nel caso in cui dai campionamenti *random* risulti una positività per la diossina, si dispongono dei controlli, questa volta a carico dell'operatore (mentre gli altri sono a carico del Servizio del Servizio sanitario nazionale, attraverso il reperimento di finanziamenti *ad hoc* nell'ambito del fondo sanitario nazionale), sulle cinque partite successive alla stessa tipologia di prodotto e di provenienza, con attivazione immediata del sistema di allerta interessati al campionamento straordinario sono in particolare i seguenti: uova e ovoprodotti, carni suine e di pollame, latte liquido e in polvere, prodotti a base di latte e prodotti a base di carne

così in altri Paesi, perché noi abbiamo già messo in atto l'etichettatura dei prodotti. Purtroppo, le *lobby* degli affari sia tedesche che di altri Paesi non vogliono accettarle in Europa, ma non vedo perché non dovremmo continuare su questa strada. Ripeto, in Italia, per quanto ne so, il problema probabilmente l'abbiamo già risolto e non dobbiamo aspettare di mettere in rete i risultati delle Regioni o aspettare i finanziamenti. Abbiamo delle forze dell'ordine, i NAS, che stanno operando bene: le posso assicurare che fanno visite in tutti gli allevamenti,

è chiaro - che lo scandalo della carne e delle uova alla diossina non era certamente un problema della sola Germania, e vorrei citare in proposito i dati della Coldiretti: «L'Italia è un forte importatore di carne di maiale dalla Germania, carne destinata soprattutto alla produzione di prosciutti (circa 13 milioni di pezzi all'anno), per un totale di 220 milioni di chili nei primi nove mesi del 2010, con un aumento del 12 per cento rispetto allo scorso anno».

L'unica certezza che abbiamo riguardo a questa legge è che ci sono due interpretazioni antitetiche: quella del giudice di Torino, che cita una sentenza della Cassazione, che avrebbe già stabilito che la norma è decaduta dallo scorso dicembre; e quella del Governo, ribadita anche alla Camera, per cui, poiché nel titolo della legge ci sono le parole «Testo unico», la norma non sarebbe toccata dal decreto taglia leggi. Non è la prima volta che questo decreto crea problemi simili. C'è dunque la necessità di fare chiarezza, ed una chiarezza massima: non sarebbe forse meglio ammettere l'errore e ricorrere ad una nota interpretativa, spiegando agli italiani il problema? Non è allarmismo questo: è chiarezza, è trasparenza. Questo è quanto chiediamo. Tutto ciò va fatto subito, perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di sapere se la loro salute è tutelata, non solo dall'attuale sistema dei controlli dei cibi, ma anche da una norma che punisca le frodi alimentari! La vicenda di cui discutiamo qui oggi, lo abbiamo detto, nasce in Germania ma è conseguenza di una situazione italiana: quella mancata tutela ambientale e del nostro settore agricolo nazionale che sta aumentando la nostra dipendenza dalle importazioni alimentari dall'estero e creando gravi conseguenze sociali, specialmente nel Meridione. Mentre oggi noi discutiamo dei problemi provenienti dalla Germania, non possiamo dimenticare che è di poche settimane fa la notizia - e lo ricordava anche lei - dell'ennesimo abbattimento di massa di capi di bestiame contaminati da diossina nella zona di Taranto. Dal 2008 1.700 i capi di bestiame che sono stati uccisi nella zona di Taranto, dove l'industria siderurgica ha inquinato irrimediabilmente le zone di pascolo. L'abbattimento di questo elevato numero di capi di bestiame contaminati è dipeso proprio dal pericolo che le loro carni venissero immesse sul mercato alimentare. Cosa sta facendo il Governo per queste drammatiche situazioni che si verificano non in Germania, non in Belgio, ma "a casa nostra", come amano sempre dire i colleghi della Lega? Cosa state facendo lei e il ministro Galan per sanare queste drammatiche situazioni e tutelare anzitutto la salute dei cittadini ed un'importantissima (forse l'unica vera) risorsa alimentare e naturale dell'Italia? Finalmente ieri la Camera dei deputati ha approvato la legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari. C'è voluto questo ultimo scandalo: non si neghi che tanti di quelli che oggi festeggiano, ieri mettevano i bastoni tra le ruote a questa legge! Da anni l'Italia dei Valori chiedeva una legge sull'etichettatura trasparente, proprio al fine di non vanificare lo sforzo di quelle imprese alimentari che investono sulla qualità e di dare ai consumatori il diritto di scelta. L'Italia dei Valori si è fatta promotrice di una simile iniziativa anche al Parlamento europeo. Certo, da Certo, da sola l'etichettatura di origine non è una misura sufficiente, in quanto appare necessario intervenire soprattutto per garantire che gli agricoltori possano continuare a produrre qualità. Ma ora tocca al Governo impegnarsi perché almeno questo provvedimento abbia effettivamente una rapida ed efficace applicazione, attraverso l'emanazione degli appositi provvedimenti attuativi. L'Italia dei Valori sarà, come sempre, vigile e pronta a segnalare se ciò non dovesse avvenire.

essere un poco orgogliosi quando vi sono dati positivi. Il sistema dei controlli, per quanto riguarda la salute dei cittadini in relazione ai ai cibi assunti, in questo nostro Paese a me pare serio e più avanzato di quello di molti Paesi europei. Io sono un convinto assertore del fatto che il futuro di questo Paese sia dentro l'Europa e sono convinto che la serietà, prima o poi, paghi. è un'antica vicenda in questo Paese, ormai quasi dimenticata per fortuna, che mise in ginocchio totalmente un settore importante della nostra produzione La serietà con la quale si lavorò per riprendersi da quella che fu una scellerata vicenda porta oggi la nostra industria enologica ad essere tra le più serie, tra le più seguite, tra le più apprezzate del mondo. Io credo che la serietà paghi: la serietà con cui ci si applica ai controlli e, in

e credo che abbia anche fatto bene, in base alla relazione che ci ha presentato, ad adottare tutti quei provvedimenti e quelle azioni politiche verso la Comunità europea.

condanne, relazioni di ordine scientifico e tecnico di magistrati e di periti dei tribunali. Noi abbiamo in Italia alcune aree totalmente inquinate.

L'unico compito forte e globale, se vuole, rimasto oggi allo Stato è quello di tutelare i livelli essenziali di assistenza. Mi dica perché in tante Regioni e in tante aree a rischio del Meridione non c'è ancora il registro tumori, molto importante. Si generano allarmismi e spesso leggiamo sui giornali che ci sono tante morti, e magari si forniscono percentuali diverse o non corrispondenti al vero. Credo

interviene su questi aspetti che riguardano l'interesse di tutti i cittadini e spesso l'interesse dei più deboli?

molto bene le potenzialità della nostra agricoltura. Credo che potremmo produrne molta di più nel nostro Paese, ma questo chiaramente è un altro tipo di ragionamento.

Questo ci fa capire oggi più che mai quanto sia importante per noi, per il nostro Paese, per tutti i cittadini e consumatori,

il valore della dieta mediterranea, che abbiamo approvato come patrimonio immateriale dell'umanità. Chiaramente l'etichettatura non fa che esaltare le caratteristiche di cui ho finora

l'allarme suscitato in Italia dallo scandalo delle uova alla diossina ci riporta alla triste realtà di come sia vulnerabile il sistema dei controlli. È necessario dotare gli alimenti di una vera e propria carta d'identità che ne riveli in qualunque momento la provenienza, gli ingredienti, il luogo di trasformazione. Tali episodi evidenziano sempre più la necessità, signor Ministro, da parte del consumatore di essere costantemente informato sull'uso consapevole di tali prodotti e tutelato da eventuali inganni, come i prodotti di alcune industrie tedesche, che spero siano punite con pene severe e certe, poiché si tratta di fatti delittuosi. Sappiamo che l'Italia è un forte importatore di maiali dalla Germania - lo ha evidenziato il collega Di Nardo - soprattutto di quelli destinati alla produzione di prosciutti. Ricordo a noi tutti che carne di maiale e salumi non contengono l'etichettatura con l'origine come le uova. Un litro di latte su cinque proviene dalla Germania e oltre alle uova anche il latte tedesco potrebbe essere stato contaminato a seguito dell'utilizzazione di mangimi alla diossina che ha portato alla chiusura di circa 4.700 allevamenti di polli e suini in Germania. Ci chiediamo quanti di questi prodotti stiano vagando per il mondo. Non possiamo sempre rincorrere le emergenze sanitarie come quella, estremamente grave, accaduta in Germania. È necessaria la trasparenza dell'informazione. Le uova ricordato il collega Vallardi - hanno un sistema di tracciabilità dal 2004, che consente di distinguere il Paese di provenienza e il metodo di allevamento. Ma io chiedo quanti di noi ne erano a conoscenza, quanti italiani sapevano come identificare le uova di provenienza italiana. La legge sulla etichettatura qui evocata da tutti e votata definitivamente da Camera e Senato fa da apripista all'Unione europea. Ricordo al collega Vallardi che questa è stata una battaglia parlamentare che è nata in quest'Aula

anche se è necessario varare una normativa europea sulla tracciabilità dei prodotti. Questa rende giustizia del lavoro e della fatica degli agricoltori e tutela la salute e la sicurezza dei consumatori. Quando è in gioco, signor Ministro, la salute dei cittadini non si può perdere tempo e cedere alle pressioni delle grandi *lobby* interessate. Bene ha fatto il Parlamento a legiferare, e bene ha fatto il Governo - gliene do atto - a mantenere quella posizione in Europa, ma ora bisogna insistere affinché l'Unione europea possa varare una normativa sulla tracciabilità. A tale proposito, insieme a tutti i colleghi del Partito Democratico, abbiamo scritto ai parlamentari europei per sostenere in Europa la tracciabilità dei prodotti. Diversamente, il nostro lavoro Ecco cosa significa maggior impegno del Parlamento e del Governo. Solo così si tutelano i prodotti alimentari e si può arginare un triste fenomeno che è tutto italiano,

La repressione, caro Ministro, oltre ad intervenire solo a valle, cioè una volta che il danno si è determinato, è effettuata con mezzi sproporzionati per difetto alla vastità delle dimensioni del problema. Il lavoro dei NAS è encomiabile, e a loro va il nostro plauso, ma non può far fronte alle incognite, specie in tempi di globalizzazione. Un accenno al tema dell'inasprimento delle pene. Ricordo subito che il ministro

decreto milleproroghe. È paradossale che l'Italia ospiti sul suo territorio l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, istituita nel 2002 a seguito di un'altra emergenza, quella della mucca pazza. se il Governo precedente ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, completamente finanziata, questo Governo si è affidato al solo ruolo, insostituibile, di repressione e controllo dei NAS e alle resistenze, è il caso di dirlo, da parte di alcuni organi ministeriali, che pongono un freno ai decreti attuativi, a differenza di ciò che hanno fatto altri Paesi europei. Ministro,

deve garantire il carattere di terzietà alla stessa valutazione. Ecco perché non comprendo la posizione del Ministero. Questo è il momento di decidere, caro Ministro. Basta giocare con la salute dei cittadini. Bene i controlli e bene l'etichettatura. Ora è il momento dell'Agenzia.

per aver ampiamente illustrato, in sette punti, quindi con una sintesi anche estremamente chiara, le azioni intraprese dal Governo in un momento di allerta internazionale che si è venuta a determinare per quanto accaduto in Germania. Il fatto che in Italia oggi abbiamo la certezza, riconosciuta anche dagli interventi dei colleghi, che tutto ciò non costituisca pericolo per i nostri consumatori è un merito che va ascritto anche alle azioni azioni di questo Governo. C'è un momento di grande serenità che, con la chiarezza che gli è propria, il Ministro ha illustrato in questo nostro incontro. Desidero esprimere apprezzamento per come sono stati tempestivamente

dei momenti di attenzione cui il Governo ha corrisposto. Tra breve mi permetterò di sottolineare in che modo. È indubbio che la tutela della produzione agroalimentare del nostro Paese è una bandiera del *made in Italy*,

ancora una volta grazie perché il Governo e il mondo sanitario si uniscono alla tutela ambientale nei momenti in cui diventa sinergico l'obiettivo della tutela dei siti dei siti di interesse nazionale. In quelle aree fortemente antropizzate, dove naturalmente anche una serie di attività alimentari o zootecniche si svolgono con i pericoli sollevati e denunciati in quest'Aula, il Governo - che interviene

l'area industriale di Taranto, diventata il simbolo negativo di una serie di problematiche connesse ai fenomeni antropici in quelle sedi. Voglio ricordare che proprio nell'area di Taranto si sono cimentati diversi Governi nazionali e regionali, ingaggiando una lotta che non ha raggiunto risultati ottimali. Probabilmente, questa sinergia tra Ministero dell'ambiente e Ministero della salute potrà creare una svolta importante anche in termini di sicurezza in quei siti. Sempre in termini di sicurezza, dopo la legge approvata definitivamente ieri alla Camera sulla tracciabilità alimentare, vorrei sottolineare che l'intervento del Governo nel Consiglio dei ministri dell'Unione europea è stato ottimale, perché ci consente di proporre, a tutela, anche qui, di quelle grandi importazioni di carni suine un momento di serenità importante. Abbiamo una nuova possibilità nel Consiglio dei ministri europeo, che richiederà naturalmente un'approvazione con i due terzi, che riconosce all'Italia

per quanto il Governo ha fatto e per quanto continuerà indubbiamente a fare in tale ambito. Questa è una politica di chiarezza e di trasparenza,

un momento di forte attenzione che porta grandi garanzie in ambito europeo e che ci rasserena. Questo è un dato per il quale intendo ringraziare il Governo ed intendo, come tutti, naturalmente, sollecitare un prosieguo di questo percorso di attenzione e di attivismo importante dell'Italia nel settore, che ci caratterizza e che naturalmente

Ritengo doveroso, come Presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, aggiungere due parole per testimoniare - come è stato fatto da tutti i colleghi di tutti i Gruppi - al ministro Fazio e al Governo

ma anche per non ingenerare quell'allarmismo che abbiamo avuto in altre epoche. Sono in Parlamento da qualche anno e ricordo crisi di interi settori e comparti della nostra agricoltura determinate proprio da allarmismi creati ingiustificatamente, a volte anche da membri del Governo. Bene, questa volta ciò non è accaduto. Questo è sicuramente un merito della serenità

con tutti i senatori di tutti i Gruppi, ha dato avvio ad una importante iniziativa legislativa che ha avuto successo, che è stata suggellata l'altro ieri da un voto positivo da parte della Camera dei deputati, e che adesso è affidata alla capacità negoziale del Ministro della salute da un lato e del Ministro dell'agricoltura dall'altro, nel consesso comunitario.

posto in Europa per la produzione di valore aggiunto e, quindi, di qualità. La norma che abbiamo prodotto tutti insieme l'altro giorno - ed è un successo straordinario per il Parlamento italiano

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro della difesa, onorevole La Russa. [LA

sul nuovo luttuoso evento che è occorso in Afghanistan, segnato dalla morte di un giovane alpino del contingente italiano impegnato nella missione ISAF e dal ferimento di un suo commilitone. Chiedo all'Assemblea di unirsi a me e al Governo per rinnovare il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari del primo caporalmaggiore Luca Sanna, che ho appena visto all'aeroporto di Ciampino, dove è arrivata la salma del militare, che stanno provando un immenso e indescrivibile dolore. Con questi sentimenti riporto il pensiero e il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale, appresa con profonda commozione la notizia, ha espresso la sua solidale partecipazione al dolore dei congiunti del militare caduto in questa missione internazionale, riportare la pace e la stabilità in Afghanistan. Rinnovo l'affettuoso augurio al militare ferito espresso dallo stesso Presidente della Repubblica. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'evento in cui ha perso tragicamente la vita il caporalmaggiore Luca Sanna è avvenuto in un avamposto della *Task Force* *North* denominato Highlander che si trova a circa due chilometri e mezzo a Est di Bala Morghab, nella provincia di Badghis, assegnata all'8° Reggimento Alpini. L'area è certamente una delle più complesse e operativamente importanti tra quelle sotto la responsabilità

12 basi italiane, di cui 11 veri e propri avamposti e una base centrale, alcune presidiate solo da italiani, altre congiuntamente con forze dell'esercito afgano e statunitense. Nell'intera area di Bala Morghab va segnalato che il numero complessivo di posizioni operative di vario tipo, anche temporanee, raggiunge il numero di 50, gran parte delle quali presidiate però da statunitensi e afgani. L'avamposto è ubicato su un'altura di circa 480 metri posta all'imbocco della valle del fiume Morghab che collega la zona alla regione del Nord. Sul fondovalle scorre l'importante strada di comunicazione denominata *Ring *Ring Road* che in quel tratto - va segnalato - è però poco più che una pista sabbiosa. Il sito Highlander ha una configurazione approssimativamente circolare, con un raggio di circa 75 metri, ed è una postazione circondata da un filo spinato, all'interno del quale vi sono diversi

In questi avamposti sono presenti due squadre di circa dieci uomini ciascuna, una italiana e una afgana. Al momento dell'evento, erano presenti nell'avamposto dieci italiani e otto afgani.

premesso, passo a descrivere gli eventi, secondo la puntuale ricostruzione che mi è stata fornita ieri (però già nei primi momenti ho avuto coerenti indicazioni) dai competenti comandi militari.

via via resa più dettagliata, ma che è rimasta assolutamente coerente con le prime informazioni. A loro va quindi il mio pieno elogio. Il 18 gennaio, alle ore 15,30, tre alpini, tre alpini, tra i quali i due poi colpiti e il caporalmaggiore Matteo Rosa, rimasto illeso, si trovavano all'aperto, protetti sul lato Ovest dell'avamposto, in prossimità del locale dormitorio (erano quindi nella parte protetta protetta dalla presenza di questo dormitorio). Trovandosi al riparo rispetto alla prevedibile provenienza della minaccia, e non essendo in servizio di guardia, stavano effettuando la manutenzione delle loro armi in dotazione, mediante l'utilizzo del compressore

comandante della postazione, e il primo caporalmaggiore Davide Frangella stavano procedendo a interventi di manutenzione sulle apparecchiature di bordo dello stesso Lince. Il restante personale era, invece, di servizio nelle postazioni che sono rivolte in direzione Est, verso l'esterno dell'avamposto.

l'afgano aveva inserito il caricatore nel fucile, cosa che non è normale se non si è di servizio, anche se non potevano sapere se l'afgano si fosse in quel momento allontanato dal servizio. Tuttavia, a voce e a gesti, gli hanno hanno intimato di estrarre il caricatore dal fucile. L'afgano ha fatto cenno di volerlo fare, ha messo la mano sul caricatore, ma anziché toglierlo, nel frattempo si è avvicinato e ha cominciato a sparare, colpendo i due militari che in quel momento non potevano reagire, poiché avevano l'arma in manutenzione e non carica, visto che non si aspettavano un attacco proditorio. Approfittando della

Gli afgani hanno provato ad inseguirlo con un mezzo lungo quella stradicciola, ma, dopo essersi diretto ad Est, l'attentatore, il terrorista, ha deviato lasciandosi scivolare nella scarpata riuscendo a eludere l'inseguimento: probabilmente era atteso o aveva previsto un modo per non farsi raggiungere. L'attentatore è stato comunque identificato come Gullab Ali Noor, nato nel Kunduz, distretto di Archi, villaggio di Sufi Zaman, in servizio da tre mesi e 45 giorni, destinato all'avamposto Highlander. Come dicevo prima, egli è riuscito comunque a fuggire nonostante la reazione degli stessi afgani e nostra. Veniva immediatamente richiesto e disposto l'intervento della squadra di reazione rapida della base di Bala Mourghab, al fine di rafforzare la necessaria cornice di sicurezza e facilitare l'intervento dei mezzi di soccorso. A scopo cautelativo veniva anche richiesto il supporto aereo, il supporto aereo, di cui però poi non vi è stata necessità. Alle 15,43, dalla vicina base Columbus, base principale dell'8° reggimento alpini a Bala partiva un'ambulanza con medico a bordo, e alle 15,46 l'elicottero Medevac statunitense. Alle 15,52, tale elicottero atterrava nell'avamposto; il medico militare verificava purtroppo che uno dei due alpini, il caporalmaggiore Luca Sanna, non dava più segni di vita. Si procedeva allora allo sgombero del caporale Luca Barisonzi che, alle ore 16,10, arrivava alla base avanzata Columbus con l'elicottero, dove veniva stabilizzato e ricoverato presso l'ospedale da campo. Nel frattempo si procedeva all'evacuazione, sempre via elicottero, della salma del militare Sanna. Alle 17,37, il ferito veniva trasportato all'ospedale Role 2 di Herat dopo uno scalo

alla schiena, alla parte cervicale, con allo stato blocco dell'utilizzo degli arti. È in questo momento in fase di decisione se l'intervento e come compierlo. Il neurochirurgo italiano ha insistito perché l'intervento venga svolto.

il 19 dicembre 2009, quando, durante le fasi di caricamento di materiali logistici su un elicottero statunitense, un militare afgano faceva partire partire raffiche incontrollate di arma da fuoco, uccidendo un soldato americano e ferendo, per fortuna leggermente in quell'occasione, due nostri militari. Per quanto riguarda la regione Ovest, di nostra responsabilità, c'è un altro episodio, che ha coinvolto però il contingente spagnolo, ancorché insistente nella medesima regione: il 29 agosto dell'anno scorso una recluta della polizia afgana esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco, causando la morte di due ufficiali e di un interprete civile, tutti spagnoli, durante un'attività di *mentoring* a favore del personale della polizia afgana in località Qal Y Naw. Addirittura in quell'occasione scaturirono disordini perché l'attentatore era uno del posto e nella confusione, dopo che egli stesso era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco di reazione da parte degli spagnoli, la popolazione aveva solidarizzato con chi credeva essere vittima e non invece carnefice. Nel quadro della ricostruzione dell'evento in cui ha perso la vita Luca Sanna, che, ricordo, era nato ad Oristano il 4 novembre del 1978 ed effettivo all'8° reggimento alpini con sede a Cividale del Friuli e coniugato (straziante oggi

colui che ha sparato aveva l'intento di uccidere, per cui non c'entra proprio niente il «fuoco amico», ma si tratta di un vero e proprio attentato, oltretutto nella maniera più subdola e proditoria,

L'evento ci fa riflettere in maniera particolare proprio perché, come abbiamo appena detto, l'azione è stata condotta da una persona che doveva essere un amico. Questo ci induce, al di là della valutazione etica e morale, a considerare che il livello di sicurezza va però adeguato anche a questa minaccia relativamente nuova, o che comunque per la prima volta ha prodotto

nel mese successivo nel Gulistan. Al momento le due aree più pericolose della zona Ovest sono, appunto, quella di Bala Mourghab, con i suoi avamposti, e le tre basi che proteggono la valle

Pensate che da noi la frequenza settimanale di eventi comunque minacciosi è pari a circa 40 (proprio in questo ultimo periodo il picco è arrivato a 40, esattamente come nella zona presidiata dai tedeschi),

è vero che la pericolosità è inferiore ma, comunque, è una pericolosità per noi elevata e a fronte della quale bisogna comunque contrapporre tutte le contromisure possibili. Quello che avevamo già rilevato è che sono diminuite

concomitanti (i mezzi tecnologicamente più raffinati che impieghiamo, i dissuasori elettronici e qualche operazione perfettamente riuscita di neutralizzazione di coloro che li fabbricavano,

non era ripresa fino adesso, quantitativamente, la minaccia attraverso attacchi suicidi che, invece, in qualche modo somiglia a quanto successo in questa occasione. Non si tratta, quindi, di mettere in discussione la bontà delle ragioni che ci portano a proseguire la missione in Afghanistan, ma di adattare e, se volete, in qualche occasione di rivedere al meglio le condizioni e le modalità di impiego dei nostri militari a fronte delle mutevoli situazioni di rischio. Quando parliamo della postazione dove abbiamo subito l'attacco, ci riferiamo migliaia di postazioni di varia natura (alcune anche temporanee) che rappresentano i sensori e gli elementi avanzati del controllo del territorio. Non possiamo, quindi, immaginare di fare a meno di questi avamposti, ma dobbiamo porci il problema di come aumentare il livello di sicurezza. dopo avere riunito i vertici militari, avevo già segnalato la mia valutazione modesta, ma che avevo pregato di tenere in considerazione, in base alla quale due settimane di permanenza in questi avamposti risultavano un periodo troppo lungo per poter mantenere alta la concentrazione e l'attenzione. Mi è stato riferito che in inverno tale permanenza viene ridotta di qualche giorno, forse anche a una settimana, ma io ritengo che, anche se il trasporto comporta altri rischi, bisogna abbassare quel livello e accrescere il nostro capo dei Servizi, il generale Santini, perché ritengo che l'*intelligence* debba svolgere un ruolo importante in questo caso e ho ricevuto l'assicurazione che, in ossequio alle indicazioni da lui avute qualche settimana fa, sono effettivamente aumentati, quantitativamente oltre che qualitativamente, gli interventi della nostra *intelligence*. Ieri, a seguito di un apposito appuntamento telefonico, ho avuto l'occasione di parlare con il generale Petraeus, al quale ho confermato l'assoluta volontà del Governo italiano e del Parlamento italiano, che si è ripetutamente espresso in questa direzione - sia la maggioranza che larga parte dell'opposizione - di tenere fede agli impegni internazionali e di non avere nessuna intenzione di scelte unilaterali. Al contempo, gli ho confermato che anche la domanda che retoricamente si è posta il Presidente è una domanda che ci poniamo tutti, ogni giorno. La vi sia un senso in questa nostra presenza. La risposta che ci diamo è che il senso c'è, ed è quello di voler mantenere vivo l'impegno farlo sarebbe un tradimento verso i soldati - di liberare l'Afghanistan e anche di mantenere forte la presenza per impedire che quel terreno diventi luogo di partenza di azioni terroristiche contro le nostre città e le nostre

a visitare il nostro contingente, non solo per rinnovare il senso di gratitudine, di stima, di apprezzamento, ma proprio per far sentire che anche l'azione del nostro Governo produce immediatamente quel *plus* di attenzione che, in casi come questi, è sicuramente

è incredibile. Nelle occasioni in cui sono andato - ero accompagnato da tanti giornalisti di tutte le testate che possono testimoniarlo - erano loro che davano coraggio, entusiasmo e forza a noi: erano loro che ci ci sottolineavano la necessità di proseguire nella loro azione. Erano loro che ci chiedevano sempre maggiore vicinanza, solidarietà e mezzi; il loro morale ci ha testimoniato come - questo è il mio convincimento - quei ragazzi e quelle ragazze facciano parte della migliore gioventù italiana. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere ancora la più profonda riconoscenza e gratitudine ad ognuno dei nostri militari e, in particolare, a coloro che come Luca Sanna sono giunti all'estremo sacrificio per garantire la sicurezza e la difesa della Patria e per la pacifica convivenza della comunità internazionale

agli obblighi che ci siamo assunti a livello internazionale nella consapevolezza dell'importanza dell'azione multinazionale per contribuire alla stabilizzazione dell'Afghanistan. Quello che non potrei mai accettare, e che credo neanche voi potreste accettare, è che eventi come questi offrano lo spunto a polemiche non solo pretestuose ma, a volte, anche legittime, che però non vorrei

Discutiamone quando volete e in ogni momento, ma diventa stucchevole, perché credo che il modo migliore per onorare quello che fanno quei ragazzi e soprattutto chi perde la vita sia quello di proseguire la loro azione o di discuterla a prescindere dal loro sacrificio. Questo è quello che ci insegna anche la dignità delle loro famiglie, da cui si trae motivo vero e profondo d'insegnamento. L'altra cosa che credo nessuno di noi voglia voglia e desideri è assistere ad un'assuefazione a questi eventi. Noi ci auguriamo che sia veramente l'ultimo, che il 2010 abbia lasciato questa coda e che non ci siano nel 2011 altri episodi luttuosi. In ogni caso, però, non dobbiamo non dobbiamo sentirci nella condizione di doverci quasi assuefare. Il fatto che l'Italia, a differenza di altre Nazioni, rinnovi ogni volta, in maniera anche istituzionale, forte forte e condivisa, la propria vicinanza, il proprio dolore e la propria solidarietà alle famiglie e a tutte le Forze armate, è per me motivo di orgoglio. Mi auguro non debbano più avvenire tali fatti, e con la stessa forza

a Roma, e magari di evitare insieme ad altre persone delle istituzioni di andare spesso, per farsi notare, una o due ore

che può fare solo con la tenacia e la forza dei nostri soldati che ci credono sul serio. Perché loro ci credono. Ecco perché partono: perché rimanere qui - le giuro - è difficile.

- non abbiamo televisione, caffè, e meno male, perché se avessimo televisioni e giornali non so come farebbero i nostri avamposti. Quindi le chiedo, signor Ministro, gentilmente di essere vicino ai nostri uomini, a tutti gli avamposti e di essere anche conscio del fatto che ci vuole un Ministro della difesa al cento per cento impegnato sul campo con i suoi uomini che le sono accanto, uomini validi, capaci (il generale Petraeus lo sa bene). Metta più *intelligence*, per favore, e quando muore uno dei nostri vorrei che almeno uno degli attentatori fosse preso.

del caporalmaggiore Luca Sanna e al giovanissimo Luca Barisonzi, che in queste ore lotta per la vita e che - come lei ci lasciato intendere - rischia di rimanere tetraplegico. Ministro, la posizione dell'Italia dei Valori è da sempre stata chiara. Abbiamo ribadito più e più volte il nostro convinto no alla permanenza delle truppe in Afghanistan. Nonostante questo, ci sentiamo comunque responsabili per quanto avvenuto l'altro ieri. Responsabili verso i genitori che hanno perso un figlio e che stanno vivendo il dramma più profondo; responsabili verso una giovane moglie che si troverà a percorrere un cammino di vita diverso da quello che aveva scelto; ma soprattutto responsabili verso quel giovane soldato che ha giurato fedeltà alla Patria e nel suo nome ha perso la vita. Ministro, nelle sue frequenti visite in Afghanistan ha mai spiegato ai nostri soldati che siamo in missione di guerra? Negli ultimi tre mesi il nostro contingente ha subito oltre 134 attacchi, di cui due con conseguenze mortali. Non ci sembrano questi i numeri di una missione di pace. Né, tanto meno, i 36 minuti di silenzio osservati dal 2001 ad oggi ci sembrano un lasso di tempo trascurabile. Questa volta, signor Ministro, gliene diamo atto, nel fornire la ricostruzione dei fatti è stato più cauto e soprattutto rispettoso dei protocolli istituzionali che è tenuto ad osservare. Ma anche ieri, comunque, non sono mancate zone d'ombra nella ricostruzione dei fatti. Emerge chiaramente una difficoltà nella comunicazione tra il suo Dicastero, quindi il suo ufficio, e le Forze armate, ma anche tra lei e il suo capo. Le vicende che hanno seguito la tragica morte del giovane alpino Matteo Miotto, il 31 dicembre scorso, ci lasciano ancora oggi senza parole. Sul decesso del militare italiano sono state date più versioni. Abbiamo assistito a comunicati tra loro contrastanti e questo è certamente poco dignitoso per il nostro Paese. È la conferma dell'incapacità di dirigere un Dicastero fondamentale come quello della difesa, come d'altronde è confermato dal fastidio dell'uscente Capo di stato maggiore della difesa. In occasione di varie interviste il generale, infatti, si è definito stupito dal fatto che lei non abbia mai cercato un confronto sulla vicenda, nonché contento dell'imminente collocamento a riposo. Tali affermazioni confermano come i problemi di comunicazione siano all'ordine del giorno e come questo recente, gravissimo episodio non sia altro che l'ultimo di una lunga serie. Ci auguriamo che lei sappia costruire col nuovo Capo di stato maggiore della difesa un rapporto migliore di quello che ha dato prova di aver instaurato con il generale Camporini. Problemi di comunicazione, Ministro, emergono anche su un altro fronte. Sarebbe forse il caso che lei e il suo capo adottaste una linea di azione comune e che non lasciaste quindi i nostri soldati, come anche le loro famiglie, di fronte a un dubbio non certo trascurabile. Le vostre reazioni a seguito dell'attentato di ieri l'altro sono state molto diverse. Lei ha affermato, dopo gli ultimi fatti luttuosi, di non aver alcuna intenzione, cito testualmente, di «mettere in discussione la bontà delle ragioni che ci portano a proseguire la missione in Afghanistan». D'altronde lo ha confermato pochi minuti fa. Al contempo, il suo Presidente si poneva un interrogativo di non poco conto e di senso diametralmente opposto, domandandosi, cito sempre testualmente, «se serve davvero restare». Lei dice che il venir meno oggi a questo impegno sarebbe un tradimento per i nostri soldati. No, Ministro, non credo proprio. Credo che questo nostro comportamento tradisca la loro dedizione. Sono controsensi che non ci stupiscono, come anche non ci sorprende il suo appoggio senza se e senza ma alla missione in Afghanistan. La sua posizione ormai sembra sempre più quella di un Ministro della guerra piuttosto che quella di un Ministro della difesa in tempo di pace. È ben nota la sua posizione guerrafondaia. Più volte l'abbiamo vista indossare la tuta mimetica e recarsi sul posto come un entusiasta giovane di leva in gita. Ha cercato persino di paragonarsi a D'Annunzio, quando, nel mese di novembre, salì su un elicottero e iniziò a lanciare sulla popolazione afgana dei volantini con messaggi di pace studiati da appositi *focus group*. Alla luce dell'ennesima disgrazia ci chiediamo se non sarebbe stato il caso di investire i soldi spesi per questa dubbia iniziativa in mezzi e sicurezza per i contingenti. Importanti polemiche a parte, vorrei porle delle domande ben precise, alle quali spero possa e sappia dare una risposta. Qual è il livello di sicurezza in cui operano i nostri ragazzi nella regione del Gulistan? Qual è il grado di collaborazione tra i nostri soldati e il neo esercito afgano? Perché siamo in un territorio che non rappresenta più ormai un covo per il terrorismo internazionale? Perché continuiamo a sostenere un Governo colluso e dedito a traffici illeciti e lontano anni luce dalla democrazia? Come mai, mentre Come mai, mentre gli Stati Uniti, a partire da luglio, inizieranno a ritirare le truppe, noi non facciamo altro che incrementarle? Sono interrogativi importanti, che mi auguro trovino risposta prima di decidere di mettere in gioco la vita di tantissimi soldati italiani. Abbiamo presentato, sia alla Camera che al Senato, una mozione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan. Concludo con una riflessione. Quest'anno ricorre il 150º anniversario dell'Unità d'Italia. Non avremmo mai voluto festeggiarlo con il nostro Paese in guerra.

Penso sia uno di quei momenti in cui le parole non riescono a trovare posto, il loro posto. È già complicato trovare il senso per le parole fuori da questi momenti, quando facciamo riferimento a questa stagione difficile in quel luogo lontano. Quante volte usiamo a sproposito il termine «guerra», raccontando magari di altre vicende, come i morti sulle autostrade o perfino gli incidenti domestici. Penso Penso che la pace - sono convinto che quella sia e resti una missione per la pace - comporti qualche volta anche i dati della guerra. Credo che sarebbe un infingimento non ragionare in questi termini, anche se a tutti noi farebbe piacere che non fosse mai necessario fare minuti di silenzio. Lei ci ha raccontato cose militari e credo che non potesse fare diversamente, perché garantire la sicurezza di quelle operazioni è un dato militare. Mi sento profondamente imbarazzato e anche profondamente inadeguato per commentare questo, pensando che forse talvolta sarebbe meglio anche per me tacere. Ma poiché questa è la dinamica del dire, dico e penso che sia giusto, come qualcuno ricordava poc'anzi, fare tutto il possibile per tempo perché quel che si può evitare si si eviti e perché ci sia il convincimento da parte di chi è lì che tutto quel che si deve fare si fa. Anch'io sono convinto che ci siano eventi nella vita per cui - come per questo accadimento, la morte di Luca Sanna - anche le parole di cordoglio a volte sembrano così difficili, forse anche così retoriche, per quanto ci si provi a trovare una modalità al massimo della sincerità possibile. Quel che è accaduto a accaduto a Luca Sanna, appunto, non può non riguardare le persone che restano, e che là restano, convinte come lei diceva che quel che fanno ha un senso.

in quel tema, in quella cifra internazionale si possono soltanto assumere decisioni. Non sono convinto che davvero farebbe bene insistere eccessivamente sulla divaricazione tra queste posizioni in questi momenti, come lei ricordava, perché ho la sensazione che questo sia il modo meno fruttuoso per dare il concreto segnale non di solidarietà di solidarietà ma di senso per chi resta. Le domande di senso ci accompagnano sempre. Figuriamoci se non accompagnano quelle persone che si vedono in prima linea, private di una intimità e di una consuetudine come è quella del lavoro con il compagno e con i commilitoni. In questo senso e con questa riflessione davvero penso che dovremmo mostrare quella responsabilità che coincide anche con l'orgoglio con l'orgoglio di sapere che ci sono ragazzi che affrontano così coraggiosamente vicende così complesse che le parole non sanno spiegare. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo parlamentare della Lega si unisce al cordoglio dell'Assemblea per questo nuovo lutto che colpisce i contingenti italiani in Afghanistan,

chiara e ci ha spiegato che gli attentati che si sono verificati hanno una metodologia diversa dal passato, il che ci deve far riflettere.

che in maniera molto chiara hanno delineato le condizioni in cui i militari operano e a quale tipo di rischi sono soggetti durante questa missione.

in maniera concreta e completa come mezzi. Il Governo non ha fatto mancare nulla, ha dato tutto quello che aveva sul territorio in termini di mezzi, mobilità, innovazione tecnologica,

un miliziano islamista riuscì a farsi esplodere in una piccola base utilizzata dai servizi segreti americani, e rimasero purtroppo uccisi 7 agenti della CIA e un loro collega giordano. La stessa cosa

Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico si associa al cordoglio di tutta l'Assemblea per la morte del caporalmaggiore Luca Sanna, si stringe attorno ai suoi familiari, che sono in questo momento in un dolore indicibile, ed esprime la più ferma e forte solidarietà per la lotta per la vita che sta conducendo l'altro militare, Luca Barisonzi,

che siamo in questo momento in un teatro di guerra. È una guerra a bassa intensità, come si dice in linguaggio tecnico, ed è certamente una guerra che per quanto riguarda la nostra presenza è pienamente dentro i limiti stabiliti dall'articolo 11 della Costituzione. Siamo infatti in Afghanistan su richiesta di un Governo legittimo e siamo lì, insieme ai nostri alleati, su preciso, chiaro, ripetuto e reiterato mandato delle Nazioni Unite.

con la serietà e la dignità necessarie, e perché questa risposta possa essere positiva mi sembra siano necessarie tre condizioni. La prima è quella di aver messo in campo una forza armata adeguata sul piano tecnico-professionale, dell'adeguatezza e sicurezza dei mezzi mezzi e del morale dei soldati, degli uomini e delle donne che rischiano la vita tutti i giorni in quel difficile contesto. Per quanto è possibile capire in Parlamento, la risposta è positiva: abbiamo avuto anche ieri un incontro importante con due alti ufficiali che hanno comandato il nostro contingente nell'ultimo periodo nell'ultimo periodo di missione e abbiamo avuto notizie confortanti su tutti e tre i fronti, naturalmente sapendo che la situazione è e resta difficile. La seconda condizione La seconda condizione è che ci sia una strategia politica chiara per l'Afghanistan a livello di alleanza e di comunità internazionale. Il contesto in Afghanistan resta difficilissimo e presenta diversi aspetti critici. Tuttavia, non si può non rilevare come la nuova amministrazione Obama, dopo una fase di riflessione, di studio, di approfondimento e anche di avvicendamento di comandanti, ha affidato al generale Petraeus obiettivi chiari, che noi condividiamo: condividiamo: rafforzamento dell'intervento per aumentare il controllo del territorio e, soprattutto, soprattutto, una rapida, intensa formazione delle forze afgane per poter arrivare poi a un avvicendamento, a una progressiva consegna della responsabilità della sicurezza sul territorio alle forze afgane, a partire da quest'anno con l'obiettivo del 2014. La terza condizione è la più importante, per certi versi la più delicata. Il fronte interno nel nostro Paese deve essere saldo perché dobbiamo essere degni, come Paese, dell'impegno e del sacrificio di questi nostri soldati. Ci deve essere un fronte interno saldo nell'opinione pubblica - e al momento vi

impegno nel collegamento tra la politica e le Forze armate. Abbiamo letto di qualche smagliatura, che ci ha preoccupato, in occasione

siamo certi che lei potrà riferirgli queste nostre preoccupazioni. Anche il comportamento del Presidente del Consiglio deve essere adeguato a questa circostanza, innanzitutto nell'esprimere dubbi e domande. Le domande e i dubbi che ha espresso ieri il Presidente del Consiglio sono domande e dubbi non solo legittimi, ma anche necessari. Vorremmo però che fossero posti nella sede giusta, che è quella della riflessione in Parlamento quando si devono rinnovare le missioni. Non è l'occasione giusta quella in cui cade un nostro soldato, perché si potrebbe insinuare il dubbio nei suoi commilitoni e nei suoi familiari

del nostro Presidente del Consiglio fosse adeguato alla circostanza nella quale si trova il nostro Paese: ventiquattro ore al giorno, di giorno e di notte. Qualche settimana fa è stata pubblicata una riflessione di un ex ambasciatore, una personalità molto autorevole della nostra diplomazia che, criticando la debolezza della politica estera italiana, diceva: l'onore dell'Italia è affidato oggi, in gran parte, al valore delle nostre missioni all'estero. Questa mattina, su tutta la stampa internazionale non si parla del nostro soldato caduto o di Bala Murghab, ma si parla di "bunga bunga";

*(PdL)*. Signor Presidente, mi unisco alle espressioni di cordoglio e di dolore per la grave perdita che l'Italia ha subito, alle espressioni di solidarietà per il ferito, che versa in gravi condizioni,

di operare nel giusto, rappresentando con onore il nostro Paese e di portare un autentico aiuto al popolo afgano.

in corso una guerra, e quindi nessuno ha il diritto di dirle che deve rendersi conto che lì si è in guerra.

perché auspichiamo, tutti auspicano, che questo esercito sia in condizioni di assumere la responsabilità e quindi di liberare i nostri da un impegno grave, difficile, oneroso. Dal punto di vista tecnico, in base alla sua esposizione, non credo si possa fare alcuna osservazione. Accetto con piacere la sua doverosa affermazione che si terrà conto anche di questo tipo di rischio e di minaccia,

proprio perché è quella più impegnata in situazioni di rischio. La solidarietà che c'è nell'ambito delle Forze armate non ha riscontro in nessun altro ente. Ma i paragoni sono sempre antipatici: diciamo che vi è una grande coesione e serietà. Allora, tutti ci chiediamo se vale veramente la pena,

anche qualche doverosa funzione pericolosa, rischiosa. È per questo che ha le Forze armate e le forze dell'ordine. Uno Stato può trovarsi coinvolto in operazioni belliche, dal momento che la guerra e le operazioni belliche esistono, sono diffuse e sono il frutto della sublimazione dell'idiozia umana. Noi cominciamo a litigare nel condominio ed arriviamo a litigare fra Stati.

È per questo che costituisce le forze dell'ordine e lo Forze armate; è per questo che combatte contro il terrorismo e la criminalità; ed è per questo che, purtroppo, a volte, perdiamo, come ha sottolineato il Ministro, i migliori della nostra gioventù. La seconda considerazione è relativa a che cos'era l'Afghanistan prima che noi andassimo lì.

allo sforzo per eliminare la più grande centrale terroristica che vi fosse al mondo, che era rappresentata dall'insediamento di Al Qaeda in Afghanistan, dalla quale erano partiti gli attacchi al cacciatorpediniere Cole, alle ambasciate di Dar es Salaam e di Nairobi, Nairobi, ed alle due Torri. Noi siamo lì perché l'Afghanistan rispose passivamente alle sollecitazioni ed alle risoluzioni delle Nazioni Unite e rappresentava una minaccia, come tuttora rappresenterebbe.

se abbiamo dei dubbi, leggiamo le lettere ed i rapporti che emergono da quanto dicevano coloro che hanno perduto la vita: sono le stesse cose che dicono i tantissimi che fortunatamente non l'hanno perduta.

Signor Presidente, a fine seduta colgo l'occasione per far presente all'Assemblea e ai colleghi un problema che sto evidenziando in questi giorni in relazione al Patto di stabilità

per cento rispetto al resto della spesa corrente, e che ha una spesa corrente di 3 milioni di euro. In teoria, applicando le norme del Patto di stabilità, nell'anno in corso, tale Comune dovrebbe accantonare, ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno, più di un terzo della spesa corrente registrata nell'ultimo anno, quindi più di un milione di euro. È comprensibile che la cosa non sia assolutamente fattibile: non è possibile cavare sangue dal muro. Come sto spiegando, non si tratta di un Comune che chieda contributi straordinari, né niente di particolare, ma solo di poter utilizzare autonomamente le risorse che ha. Credo che dobbiamo assolutamente dare risposta a questo tipo di esigenza, trovando delle norme che non vadano a ledere l'autonomia degli enti locali e che, allo stesso tempo, li carichino ovviamente della giusta responsabilità.

dei *crack* finanziari sistemici, ha ridotto purtroppo gli utili, per cui anche i dipendenti, ossia i poveri commessi,

ai Governi, alla loro solvibilità e con i loro rapporti influenzano anche le speculazioni di Borsa sui mercati, sulle azioni, sulle obbligazioni e sui titoli di Stato. Il 6 maggio scorso

di sottolineare che il tema di questi Comuni, e in special modo di alcuni Comuni veneti, che si sono venuti a trovare in questa particolarissima situazione è all'attenzione di tutti,

senza mettere mano all'impianto complessivo del Patto di stabilità che, come tutti sappiamo, ci chiama ad assumere impegni che non dipendono solo da noi, ma che stanno nell'equilibrio della nuova *governance* economica europea.

e testi bancari che regolano la vita delle nostre banche, delle nostre società finanziarie e dei vari istituti che a vario titolo, come anche i fondi d'investimento, operano su un fronte delicatissimo come quello del risparmio gestito, sia arrivato forse il momento di aprire una riflessione più ampia (a freddo rispetto alla crisi datata due anni fa, ma ancora sufficientemente a caldo per vederne tutti gli effetti negativi anche nel nostro sistema Paese) insieme insieme al Governo, in un *continuum* tra Parlamento e Governo, su un tema di così rilevante importanza, perché si proceda per gradi, ma complessivamente e in modo unitario, a una riforma della legge bancaria italiana: dalle banche popolari alle fondazioni, ai fondi d'investimento, al risparmio gestito. Una nuova legge bancaria che aggiorni, alla luce di quanto accaduto nel resto del mondo, ma anche nel nostro Paese in questi ultimi anni, e che ci consenta di accompagnare il sistema bancario e finanziario, così importante, gamba fondamentale del sistema economico e del sistema Paese, in un processo di modernizzazione e di evoluzione nella direzione della trasparenza, dell'efficienza e dei minori costi che devono poi ricadere sui risparmiatori, che sono la linfa vitale di questo Paese. Se il nostro Paese ha potuto affrontare questa crisi, non dimentichiamolo mai, lo ha potuto fare in virtù di un risparmio privato elevatissimo, gli consente di avere garanzie sufficienti per potere ogni mattina, quando si apre la Borsa, resistere alle intemperie dei mercati finanziari.